Presidente, avendo raggiunto già l’accordo unanime in Commissione, non credo ci siano grossi problemi. Con l’Accordo al nostro esame tra Italia e Kosovo ci si prefigge l’obiettivo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia per contrastare la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo internazionale. È lo strumento giuridico, quindi il contorno, per regolamentare la collaborazione operativa tra le varie forze di polizia. Esso definisce le autorità competenti per l’Italia è il Ministero dell’interno - e i settori di cooperazione, quali la criminalità informatica, il traffico d’armi, i reati economico-finanziari e il traffico di stupefacenti. Prevede anche delle riunioni periodiche nei vari Stati, tra le forze di polizia, e disciplina lo scambio di informazioni, anche classificate. Lo riteniamo un Accordo molto utile, soprattutto in questo periodo e, visti i recenti eventi

firmato tre anni fa con un Paese che ha ancora bisogno di attenzione e di accompagnamento, in un processo di stabilizzazione dei Balcani e in una prospettiva di avvicinamento alle istituzioni europee; in un territorio dove ancora, nel Nord, ci sono problemi di convivenza fra la comunità di etnia albanese e quella serba e dove si sono svolte le elezioni municipali con una partecipazione intorno al 10 per cento, boicottate dalla comunità serba e con alcune tensioni. C’è quindi la necessità di un accompagnamento dei Paesi europei, in particolare dell’Italia, che è sempre stata presente, in un’ottica di stabilizzazione e di sicurezza per garantire la convivenza fra i popoli. Un Accordo di questo genere è sul modello di altri già conclusi, in cui la nostra forza di a costruire istituzioni democratiche e a formare corpi dedicati alla tutela dell’ordine pubblico e a garantire la sicurezza soprattutto in quella parte di territori dove le tensioni in questi anni sono state più forti. Quindi, il nostro non può che essere un voto favorevole.

Signor Presidente, alla luce di quanto dichiarato ieri in discussione generale, considerando la lotta alla criminalità organizzata come una priorità da perseguire,

Sappiamo che si tratta di contesti nei quali spesso ci sono ancora fasi molto impegnative, per cui l’intervento legislativo

esprime a favore anche degli Accordi che esamineremo successivamente e che riguardano la materia radiotelevisiva nell’Accordo tra la Repubblica italiana e San Marino (un antico Accordo del 2008 che viene rinnovato) e la ratifica

Grazie.

in questione prevede un quadro giuridico per incrementare i rapporti su molti aspetti del vivere comune, se sia possibile avere un report del Ministero degli affari esteri

prevedere o rivedere eventualmente detti accordi in modo che vengano utilizzati dalle nostre industrie, dalle nostre università e da tutti i nostri attori istituzionali. Per tali ragioni esprimo un voto favorevole anche sul citato Accordo.

Signor Presidente, nell’annunciare il voto favore- vole a questa ratifica, esprimo grande soddisfazione, essendo stata io sindaco di Coriano, primo Comune di confine con la Repubblica di San Marino, in quanto si conferma anche qui in Senato un rapporto di collaborazione proficua tra i due Stati.

(PD-IDP). Signor Presidente, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, a mia prima firma, ha lo scopo di ratificare l’Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Costa Rica, firmato il 27 maggio del 2016. Le relazioni bilaterali - come credo di aver detto ieri in discussione generale - tra questi due Paesi sono ottime, solide e improntate ad un fiducioso rapporto di amicizia e collaborazione. L’ottimo andamento delle relazioni bilaterali è anche confermato dalla piena collaborazione, soprattutto nei fori multilaterali, con numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. 6 Settembre 2023 della Costa Rica alla candidatura italiana al Consiglio di sicurezza dell’ONU cinque anni fa. Inoltre, tali relazioni sono favorite dai soliti rapporti commerciali fra i due Paesi. La Costa Rica è, infatti, il quarto più importante partner dell’Italia nell’area dell’America centrale dopo Messico, Panama e Cuba, con un interscambio globale che solo nel 2015, quindi l’anno prima della firma, ha raggiunto la cifra record di 379,5 milioni di euro. Questo Accordo si inserisce quindi nel contesto di un rilancio delle relazioni bilaterali dell’Italia con uno dei partner tradizionali storici dell’America centrale, un Paese che si caratterizza per la grande stabilità politica, una delle più elevate dell’area. Non è mai stato firmato prima uno specifico accordo nel settore perché esisteva un accordo quadro tra Italia e Costa Rica firmato nel 1983, riguardante principalmente la cooperazione economica, finanziaria, sociale e culturale. L’Accordo si compone di 21 articoli. Gli articoli da 1 a 3 definiscono l’impegno delle parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati; a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture

che gli articoli da 6 a 8 rappresentano uno degli aspetti più interessanti dell’Accordo, avendo come scopo il rafforzamento della collaborazione nel campo dell’istruzione mediante lo scambio di esperti, informazioni e documentazione, anche al fine di riconoscimento ed equiparazione dei titoli universitari. Signor Presidente, La Costa Rica è uno dei Paesi della mia circoscrizione elettorale. Come già detto, alcuni mesi fa ho avuto il piacere e l’onore di visitare e conoscere meglio questo Paese e personalmente molti membri della storica e operosa comunità italiana che ha dato un sostanziale contributo allo sviluppo del Paese, oltre ai tanti giovani imprenditori che vi risiedono. Nei miei contatti diretti con la collettività italiana - un numero che in realtà aumenta ogni singolo anno - ho potuto riscontrare personalmente quanto sia auspicata la ratifica di questo Accordo, non soltanto dagli oltre 6.000 iscritti all’AIRE che vivono in Costa Rica, ma anche e soprattutto da migliaia di altri cittadini italiani residenti in quel Paese e anche dai non iscritti all’AIRE, e per i costaricani che vivono in Italia, nonché per tutte le istituzioni culturali e scientifiche. Per queste ragioni, Presidente, comunico il mio pieno appoggio e il mio voto favorevole alla ratifica di tale Accordo.

i contenuti dell’Accordo di cui si chiede oggi la ratifica all’Assemblea, annuncio e confermo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d’Italia.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 28 settembre. La prossima settimana sarà discusso il disegno di legge di delega al Governo per la revisione degli incentivi alle imprese, collegato alla manovra di finanza pubblica. Gli emendamenti al provvedimento - con le modalità di cui all’articolo 126-bis del Regolamento - dovranno essere presentati entro le ore 12 di lunedì 11 settembre. Il calendario prevede inoltre la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge su diagnosi e prevenzione del diabete di tipo 1 e della celiachia, approvato dalla Camera dei deputati. Nella giornata di mercoledì 13 settembre saranno discusse mozioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella settimana dal 19 al 21 settembre saranno discussi, dalla sede redigente, i disegni di legge su iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe e sull’istituzione dei nuovi giochi della gioventù. Mercoledì 20 settembre, alle ore 10, saranno esaminati documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Il calendario della settimana dal 26 al 28 settembre prevede la discussione del decreto-legge sugli investimenti strategici e del decreto-legge - attualmente all’esame della Camera dei deputati - in materia di processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, personale della magistratura, salute e cultura. Giovedì 14, 21 e 28 settembre avranno luogo il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il question time. Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge di disciplina della professione di guida turistica, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Conferenza dei Capigruppo, ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento, il Gruppo MoVimento 5 Stelle fa proprio l’Atto Senato 127, a prima firma del senatore Turco, avendo avuto il numero sufficiente di firme.

Dopo le notizie degli spaventosi abusi perpetrati per mesi a Caivano da un gruppo di almeno una quindicina di ragazzi giovanissimi su due bambine di dieci e dodici anni, pochi giorni fa un altro atroce episodio si è verificato in pieno centro a Napoli,

Non è stata Caivano a stuprare e non è stata Napoli ad ammazzare: il mandante occulto è lo Stato, che ha clamorosamente fallito, lasciando i propri cittadini in balia di un ordine sociale gestito dalla cultura della violenza, della barbarie e della prevaricazione. Infatti, dove lo Stato non c’è, imperano e governano le mafie. Onorevoli colleghi e colleghe, smettiamo di chiamarla emergenza: questa è una situazione radicata, endemica; è un abisso senza fondo, per il quale non si è fatto e non si fa nulla. Interi quartieri e migliaia e migliaia di ragazzi lasciati a loro stessi, con tassi di abbandono scolastico che toccano picchi del 34 mancanza di alternative sane e di prospettive lavorative, impigliati nelle reti criminali e in balia di sguardi vuoti, voltati altrove, nella completa indifferenza di tutti. assenza dello Stato diventa addirittura accanimento nelle Regioni del Centro Sud. Penso alla revisione del Titolo V della Costituzione, che ha innescato un progressivo disinvestimento nelle scuole centro-meridionali e alla mancata applicazione della clausola del 34 per come confermato da Eurispes, ha sottratto al Sud 840 miliardi di euro netti a cavallo tra il 2000 e il 2017. Questo per non parlare delle conseguenze della folle deriva dell’autonomia differenziata nei territori fragili del Paese: è qui che c’è la povertà e che prospera la delinquenza; anzi, la povertà è correlata indissolubilmente alla delinquenza. Si sta tanto parlando di bonifica e di estirpazione: queste sono le parole pronunciate dalla presidente Meloni, che sono davvero aberranti, i terreni e le paludi si bonificano ma le persone si educano. All’indomani dell’omicidio del povero musicista, ho sentito a un TG le parole del direttore artistico della Nuova Orchestra Scarlatti, che ho avuto il piacere di sentire poco prima dell’estate: se ci fosse stata un’orchestra stabile a Napoli in questi anni - ha ammonito il maestro Gaetano Russo - il ragazzo ucciso non sarebbe stato lì, ad arrotondare come cameriere. Come dargli torto? E qui mi rivolgo al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, affinché accolga il suo appello. Onorevoli colleghi e colleghe, probabilmente se il killer - perché il ragazzo che ha sparato si è comportato da vero killer - fosse stato educato in un contesto culturale differente, probabilmente a quell’ora non sarebbe stato sveglio e non avrebbe impugnato la pistola. chi gli ha procurato la pistola era un maggiorenne. Mi chiedo inoltre: erano lì per uccidere qualcuno? E ancora mi chiedo: se gli stupratori fossero cresciuti in un contesto culturale differente, ben lontano da logiche deviate di abbandono sociale, forse non saremmo qui a parlare di Caivano. La storia però non si fa con i se e con i forse, ma si cambia con i fatti concreti forse, ma si cambia con i fatti concreti e qui l’unica vera rivoluzione che si deve innescare è di tipo culturale, scolastica ed educativa, cioè prevenire, investendo nella scuola. Grandi economisti hanno affermato che con un euro investito nella scuola se ne producono 2,5. La scuola prepara i cittadini e li rende consapevoli di sé, pronti a essere inseriti nel mondo del lavoro. Questo è il vero grimaldello con cui scardinare la povertà, la malavita e il disagio sociale.

Signor Presidente, nella notte tra il 5 e il 6 settembre di tre anni fa, a Colleferro veniva massacrato di botte e ucciso Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di origine capoverdiana che viveva a Paliano con la sorella e i genitori, cuoco nel ristorante di un hotel poco distante.

storia di coraggio e di improvvisa e inaudita violenza ha colpito tutto il Paese. Il suo sorriso, che non stinge sui muri, si va a sommare agli altri mille volti di vite interrotte dall’odio, dalla ferocia e dalla rabbia che si agita, Presidente, sulla superficie di questo nostro Paese e delle sue città come Colleferro, faticano con dignità e difficoltà a trovare una loro missione e a cucirsi in una comunità che sappia assorbire questo dolore e che, nonostante tutto, sappia farlo fiorire senza che appassisca nella vuota illusione del «mai più» delle celebrazioni. come ogni giorno, a Colleferro si ricorderà Willy, ci si riunirà in suo nome, con una presenza nel ricordare che è anche soffrire di nuovo la sua quotidiana assenza. È uscito un libro necessario di Christian Raimo e Alessandro Coltré su questa storia di ragazzi. Aurelio Picca ha girato un documentario, «Preghiera per Willy», partendo proprio dal luogo dell’assassinio spietato che oggi, Presidente, diventerà finalmente una piazza,

è destinato il futuro. Ecco, Presidente, io non lo so: di solito, all’innocenza è destinato il suo passare, il suo mutarsi nel suo rovescio, che non è l’esperienza o la condizione adulta e neanche il corrompersi, ma il non esserci più, l’immanenza che scolorisce, perde vigore, invecchia e muore. di Willy Monteiro non è stato dato il tempo di trasformarsi nel suo tramontare. Per questo, Presidente, il suo trauma, avvenuto nell’anno del Covid, è collettivo e richiede uno sforzo di racconto, di comprensione, di lutto e di responsabilità collettiva, cosa che la sua città proverà di nuovo a fare oggi e che noi qui in quest’Aula offriamo oggi come devozione, per la sua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

con il seguente ordine del giorno: I. Discussione dei disegni di legge: Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese (607) (voto finale con la presenza del numero legale) - Relatore PAROLI PAROLI II. Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge: Deputati MULE’ e Laura CAVANDOLI. - Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica (approvato dalla Camera dei deputati)

Grazie.